nel corso della seduta. senatori, desidero rivolgere un commosso pensiero di vicinanza e cordoglio ai familiari, ai colleghi e agli amici della senatrice Emilia Grazia De Biasi. Donna di brillante intelligenza e inesauribile energia, Emilia De Biasi è stata un'autentica protagonista della vita politica nazionale degli ultimi anni. Consigliere comunale a Milano, sua città di adozione, deputata per due mandati, dal 2006 al 2013 e, quindi, senatrice della XVII legislatura, Emilia De Biasi ha sempre interpretato il suo ruolo all'interno delle Istituzioni con grande coerenza e con grande concretezza. Come Presidente della Commissione igiene e sanità del Senato seppe raccogliere la stima e l'apprezzamento di tutti i colleghi per l'imparzialità e l'autorevolezza dimostrate in ogni occasione, insieme alla sua costante apertura al confronto costruttivo. Un carattere forte e determinato, il suo, ma anche profondamente umano e sensibile alle tante difficoltà quotidiane di chi è più debole o versa in situazioni di particolare fragilità. Quello stesso carattere che l'ha sostenuta e guidata in tante iniziative e tanti progetti intrapresi, dentro e fuori dalle Aule parlamentari, per promuovere e difendere la parità di genere, il diritto alla salute e la cultura come strumenti insostituibili di crescita umana e progresso sociale. Con Emilia De Biasi ci lascia una politica appassionata, una donna coraggiosa e intraprendente, che non ha mai smesso di battersi per quegli ideali di libertà e dignità umana in cui fortemente credeva. Ricordarne la figura e il suo instancabile impegno civile e politico, significa soprattutto tenere viva la memoria di un esempio di vita dedicata ai valori di una democrazia matura, dialogante e responsabile, così come alla volontà di lavorare bene sempre e comunque nell'interesse superiore dei cittadini. In ricordo della senatrice Emilia Grazia De Biasi, invito pertanto l'Assemblea ad osservare un minuto di silenzio.

appena pronunciato e per il ricordo di Emilia. Molti in quest'Aula l'hanno conosciuta durante la scorsa legislatura e hanno potuto riconoscere in lei una donna non comune, intelligente, determinata, lavoratrice appassionata. Emilia era una donna libera, gelosa della propria libertà. Amava formarsi le opinioni studiando, leggendo e, se era necessario, non aveva timore a esprimere opinioni non scontate, a volte scomode, che sosteneva in modo appassionato, anche rischiando di andare sopra le righe. Emilia era una donna libera, colta, non comune, che ha dedicato la sua vita e i suoi talenti alla politica, alla difesa della Costituzione, ma prima di tutto alla sua città, Milano, di cui è stata consigliere comunale e che è sempre stata al centro della sua attività politica e parlamentare. Accanto a Milano per Emilia c'era l'elaborazione delle politiche femminili, che è stato il filo conduttore che ha segnato la sua vita e su cui ci ha lasciato tanto.

per sostenere la cultura e rendere fruibile a tutte e a tutti quella cosa, Emilia capiva davvero di cultura, di musica e di teatro: su questo aveva tanto da insegnare e questa sua sensibilità le ha dato la possibilità di coltivare tante relazioni e di entrare in rapporto con mondi spesso lontani dalla politica. In questo ramo del Parlamento Emilia ha lavorato poi per un'intera legislatura come Presidente della Commissione sanità: ha fatto mentre si discutevano temi importanti e controversi. Tenne una posizione difficile, ma coerente e alla fine vincente, sulla vicenda di Stamina: lo fece con coraggio, sfidando le minacce odiose che le arrivarono. Con la stessa determinazione si espose ai no vax e sostenne la legge Lorenzin. Chi l'ha conosciuta non può non aver ricordato in questi giorni, in cui la questione delle vaccinazioni diventa centrale per sconfiggere la pandemia, il suo impegno su questo. Emilia De Biasi ci ha abbandonato presto, troppo presto, ma non ha mai perso un minuto della sua vita per migliorarsi e guardare il mondo. L'ultima volta che ci siamo sentiti era entusiasta, mentre aspettava di iniziare un nuovo ciclo di chemioterapia, perché la sua vista era migliorata e finalmente riusciva a leggere. Emilia era così, amava soprattutto alimentare il pensiero e le conoscenze. A nome del Gruppo Partito Democratico voglio esprimere a Guglielmo, suo marito, alla mamma e ai fratelli la nostra vicinanza e le condoglianze, dicendo loro che che siamo orgogliosi di aver lavorato con lei e che le tante cose che ha fatto e ci ha insegnato la faranno restare con noi.

ho conosciuto la senatrice Emilia De Biasi all'inizio della scorsa legislatura, in occasione dell'insediamento della Commissione sanità di cui facevo parte e della quale diventò presidente. Sin da subito ebbi la sensazione che il presidente De Biasi fosse una persona estremamente gentile e disponibile, ma dal carattere molto determinato, a tratti sanguigno e autenticamente interessata a preservare e possibilmente migliorare il nostro Sistema sanitario nazionale nella sua universalità ed equità. Emilia De Biasi era anche un'appassionata della Valle d'Aosta. Per alcuni anni ha frequentato il Comune di Gaby nella valle di Gressoney in quelle occasioni ho avuto il piacere di accompagnarla a visitare le strutture socio-sanitarie della mia Regione, dimostrando lei sempre una grande attenzione all'erogazione dei servizi nei territori, e di ospitarla anche in occasione di convegni ai quali partecipava con competenza e passione. Ricordo che, quando ci si incontrava qui in Senato, mi salutava con un «*Bonjour, monsieur le sénateur*», come vengo chiamato dalle mie parti, con un R rotante che rendeva il francese ineccepibile. Vorrei brevemente ricordare quanto furono determinanti la sua azione politica e il suo ruolo di presidente della Commissione sanità nel rendere possibile l'approvazione di leggi importanti come quella sul riordino delle professioni sanitarie, quella contenente disposizioni in materia di sicurezza delle cure per i cittadini, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie. Ricordo anche la legge quadro sui disturbi dello spettro autistico e l'approvazione - l'ha già ricordato il collega Mirabelli - della legge sui vaccini, con la grande battaglia sulle vaccinazioni che ho avuto l'onore di condurre anche al suo fianco. Guarda caso, un tema attualissimo. Ricordo ancora molto bene la passione e la competenza dei suoi interventi in Aula. Cara Emilia, grazie per tutte queste battaglie e per il tuo impegno per una società più giusta a sostegno, in particolare, dei diritti delle donne e dei più deboli e, soprattutto, grazie per la tua amicizia. Riposa in pace.

Signor Presidente, Emilia De Biasi era una donna colta e di grande spessore intellettuale. Ricordo che una sera, dopo faticosissimi lavori in Aula, mi trascinò dall'altra parte di Roma per assistere a uno spettacolo di sperimentazione teatrale. Pioveva a dirotto, ma lei caparbiamente mi trascinò lì. Con lei si parlava di libri, cinema, teatro e viaggi. Questa appassionata curiosità per la vita Emilia De Biasi la trasferiva nel suo impegno politico. A volte, esprimeva disagio per le nostre comunità politiche - chi non ha momenti di difficoltà? ma andava sempre avanti. Era sempre propositiva e fiduciosa nel voler cambiare e trasformare il mondo in meglio e riportare il bisogno di relazioni umane in politica. Anche in queste ultime settimane ne parlavamo. Da parlamentare e da Presidente della Commissione igiene e sanità per cinque anni - è stato ricordato - il suo impegno è stato per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria. Il testo è diventato legge. Si è impegnata sulla responsabilità professionale del personale sanitario sulle disposizioni anticipate di trattamento. Lei era relatrice e si dovette dimettere con sofferenza per agevolare il percorso. La legge fu approvata. Sul provvedimento sui vaccini - è stato ricordato - in prima lettura sono stati apportati cambiamenti al testo grazie a un'approfondita istruttoria svolta dalla Commissione. Il decreto è stato convertito in legge. Ricordiamo il suo impegno sull'inquinamento ambientale legato alla salute e alla possibilità di ammalarsi di tumore. Se vogliamo prendere un filo conduttore della sua Presidenza, possiamo parlare di un dialogo tra scienza e politica (in quegli anni emblematico fu il caso Stamina). Ma adesso, ancora oggi, questo tema è fondamentale: scienza e politica. poi una questione che sembrerà banale: la Commissione intera affrontava un affare assegnato sul superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari. Noi, la Commissione igiene e sanità l'aspettavamo per un'audizione nell'ambito di un affare assegnato sulla medicina territoriale, come presidente di All.Can Italia, il suo ultimo impegno, sull'oncologia di prossimità. Lei diceva che noi dobbiamo concepire il paziente al centro dell'innovazione, proprio perché sempre attenta alle innovazioni, con una curiosità straordinaria. Il presidente De Biase non verrà in audizione, ma di una cosa siamo certi: ci consegna un compito arduo, continuare il suo impegno competente e appassionato per la cultura, le donne, la salute e il bene comune del nostro Paese. Soprattutto, per chi ha avuto il dono di conoscerla, ricordo la sua profonda umanità, anche espressa con una risata, con una voce dolce e altisonante allo stesso tempo. Questa sua profonda umanità dovrà contagiare tutti noi nel nostro impegno civile, perché la ricordiamo sempre lì, fuori e dentro le Aule, con questo suo atteggiamento profondamente umano e competente. Quanto ha insegnato, nella passata legislatura, a noi nostra prima legislatura; quanto ci ha insegnato, anche con una generosità minima, anche nei piccoli gesti, anche comportandosi in un certo modo, per l'attaccamento istituzionale. Alla sua famiglia anch'io esprimo, a nome del Gruppo Italia Viva, Viva, profonde condoglianze, al suo amato marito e a tutti quelli che l'hanno conosciuta.

doloroso ricordare Emilia, non solo perché stiamo parlando di una persona cara che non c'è più, perché, per quanto mi riguarda, il ricordo di Emilia fa vivere in me il ricordo di una militanza e di un percorso comuni, che sono stati importanti e fondamentali nella mia biografia politica. Ho conosciuto Emilia molti anni fa e questa conoscenza si è dispiegata in uno schema, se volete, classico e tradizionale (o almeno lo era nelle antiche comunità politiche), cioè in un rapporto tra esponenti

lunga esperienza politica, sul territorio e anche a livello nazionale. Però lei era attraversata dalla consapevolezza che una delle funzioni delle comunità politiche e dei partiti dovesse essere quella di individuare e selezionare la classe dirigente e di farla crescere, in un rapporto tra generazioni che doveva essere franco e dialettico. Lo dico con un sorriso, perché chi conosce Emilia sa sa cosa voglia dire avere un rapporto dialettico con lei (usando naturalmente un eufemismo). Tale rapporto era sempre incentrato sulla consapevolezza che le classi dirigenti non cascano dal cielo, ma sono il frutto di una costruzione paziente e costante, di un rapporto e di un confronto, anche tra tra esponenti di generazioni diverse e di percorsi diversi. Io devo molto a Emilia anche da questo punto di vista. Lo hanno ricordato i colleghi che mi hanno preceduto: Emilia era una donna coraggiosa e determinata, che ha informato la sua lunga esperienza politica non solo a una tesi che io condivido (il legame profondo tra la sfera dei diritti civili e i diritti sociali), ma anche alla profonda convinzione che la attraversava che gli stessi diritti civili, di cui lei si è occupata da sempre, avessero anzitutto la caratteristica della loro indissolubilità. pensava che non ci fossero le battaglie delle donne, le battaglie per i diritti LGBT, le battaglie per l'infanzia, le battaglie per le fragilità, ma che ogni battaglia vivesse della forza delle battaglie per gli altri e che rafforzare i diritti di ciascuno volesse dire rafforzare i diritti di tutti gli altri. Questo era il suo pensiero, questa era la sua convinzione io credo che il debito che abbiamo con una personalità, con una figura come quella di Emilia sia esattamente questo: comprendere, nel mondo nuovo nel quale stiamo entrando, l'importanza di una riflessione di questo genere, che lei naturalmente faceva vivere nell'esercizio della sua funzione parlamentare e nella sua iniziativa politica. Grazie in ragione della competenza che lei ha acquisito nel corso di tanti anni, soprattutto sul tema non tanto della salute, che può sembrare un riferimento settoriale, ma sul tema della cura

la sua competenza proprio nella fase difficile che stiamo vivendo ci mancheranno. Ci mancheranno anche quel sorriso e quella risata travolgente che si faceva notare Grazie Emilia, ci mancherai molto. Grazie È con grande rammarico per la sua scomparsa e con commozione che ricordo la senatrice De Biasi. Ebbi l'onore di essere Vice Presidente, nella scorsa legislatura, quando lei era Presidente della Commissione sanità. Insieme facemmo molte battaglie, battaglie vere, a volte ovviamente anche per differenze di opinione. Ricordo, sulle disposizioni anticipate di trattamento, quando io insistevo perché fosse lasciata ai medici la libertà di coscienza. Ricorderò sempre una frase di Emilia: «Donne, cultura, informazione, lavoro». Queste sono le quattro parole che ho nel cuore e che difendeva senza paura di fronte a nessuno. Agli inizi, nella nostra Commissione, a volte eravamo un po' allibiti, perché Emilia era una donna molto spontanea e spesso la sua veemenza ci lasciava un po' interdetti, ma imparammo prestissimo a conoscerla, a conoscerci e ad apprezzarci. Lei era una donna vera, non conosceva l'ipocrisia, si poteva capire il suo pensiero dal suo volto. Ho ancora presente l'immagine di quando, magari dissentendo dagli interventi di qualcuno di noi, alzava gli occhi al cielo o inarcava il sopracciglio e poi sapevo che il mio compito era sempre quello, passato il temporale, di fare in qualche modo da pompiere. Sentiva la Commissione sanità come una famiglia e ricopriva questo suo ruolo di Presidente con grande orgoglio. Ricordo un giorno, quando in audizione proprio a proposito del decreto Lorenzin c'era un audito che rappresentava i no vax e che insultò tutti noi commissari, dandoci degli ignoranti e dei venduti il presidente De Biasi lo interruppe di colpo e lo fece immediatamente uscire dalla Commissione. Molte cose portammo avanti in quella legislatura, argomenti importanti, come appunto quello sulle disposizioni anticipate di trattamento, la legge sui vaccini, che è stata ricordata; dopo vent'anni si riuscì a portare a termine la legge per il riordino delle professioni sanitarie, si portò a termine anche la legge Gelli sulla responsabilità civile dei medici, che però non è ancora molto utilizzata, visto che mancano, a distanza di quattro anni, i decreti attuativi. Si fece un'indagine conoscitiva molto accurata sulla sostenibilità del sistema sanitario. I risultati di questo documento sono ancora oggi - anzi, soprattutto oggi - attualissimi. Per questo Emilia ricevette anche un premio dalla fondazione GIMBE per il suo impegno

disse: quante donne, anche giovani, avremmo potuto curare per tempo se gli ospedali nelle diverse Regioni avessero fatto quello che dovevano fare, cioè informare i cittadini e consentire alle donne di decidere, con loro e per loro, percorsi diagnostici e di prevenzione a partire dagli *screening*? Questo purtroppo non viene fatto e lo sappiamo perfettamente. Non possiamo tollerare che le capacità professionali di tanti medici vengano umiliate nel non poter curare le donne perché ci sono scelte che decidono di andare in un'altra direzione e spendere i soldi della prevenzione, per altro, se non addirittura, con gravi problemi anche di legalità. *(Applausi)*. Credo che su questo dobbiamo fare uno sforzo, dando pari opportunità alle donne nel campo della salute.

non può mancare anche il mio ricordo in questo momento ripensando a Emilia De Biasi. Ho avuto l'occasione e l'onore di essere insieme a lei in XVI legislatura in 7ª Commissione,

e l'amore che traspariva anche dalla trattazione dei vari provvedimenti; un amore grande per la cultura in qualunque sua forma, che fosse la musica, i libri, l'editoria il suo *blog* sul rock. Era veramente poliedrica, con un entusiasmo straordinario e una voglia di vivere tutti i momenti

presente sempre anch'io: abbiamo vissuto cinque anni insieme, tutti i santi giorni, in Commissione. È stato un rapporto costruttivo perché, come è già stato detto, Emilia amava anche il confronto

che con Emilia perdono non solo un'amica, ma un componente fondamentale, per come ha voluto vivere la sua passione politica,

la senatrice De Biasi, scomparsa davvero prematuramente, era originaria del mio territorio, essendo nata a San Severo, in provincia di Foggia, ma era milanese d'adozione, come è stato ricordato più volte.

Il suo impegno politico si è esplicitato su più fronti. Diceva infatti: «Donne, cultura, informazione e lavoro sono le quattro parole che ho a cuore» infatti la sua azione è stata sempre rivolta alla difesa delle donne, dei loro diritti, della parità di genere in ogni ambito, sia in famiglia, che nel lavoro, nel sociale e nella vita politica. Nell'ambito culturale il suo apporto è stato tangibile, come dimostrano l'approvazione della legge sullo spettacolo dal vivo, ma anche la legge sull'equo compenso ai giornalisti autonomi, la riforma dell'editoria, le misure di agevolazione fiscale per il cinema e per il riconoscimento dell'indennità di disoccupazione per gli artisti. Come hanno ricordati i colleghi, è stata Presidente della Commissione igiene e sanità del Senato nella scorsa legislatura e anche in questo campo ha dato il suo fattivo e concreto contributo, lavorando perché si arrivasse ad importanti progressi di civiltà e di rispetto della dignità dei pazienti. Mi riferisco in particolare alle disposizioni anticipate di trattamento, un tema che che in Italia rientra in un ambito sempre particolarmente delicato, al consenso informato e alla responsabilità degli esercenti la professione sanitaria. anche impegnata per l'approvazione della riforma degli ordini e delle professioni nell'ambito della salute, per il rafforzamento e l'ammodernamento del Servizio sanitario nazionale, per garantire la sua universalità ed equità, specialmente nei confronti delle categorie più fragili. Si può affermare con sicurezza che ha sempre lavorato per la valorizzazione di quello che potremmo definire il capitale umano del nostro Servizio sanitario nazionale e per promuovere il dialogo e il confronto tra le istituzioni e le organizzazioni dei cittadini e dei pazienti. Proprio grazie a questo suo impegno indefesso nel comparto della salute ha ricevuto, nell'anno 2016, dalla fondazione GIMBE, il riconoscimento intitolato «Salviamo il nostro Servizio sanitario nazionale». Alcune scelte ci hanno diviso, come è normale e come succede in politica, ma posso affermare con sicurezza che, con la scomparsa di Emilia De Biasi, perdiamo una donna che ha dedicato la sua vita agli altri e alla politica, sempre attenta ai bisogni dei cittadini e al rispetto e al rafforzamento delle istituzioni repubblicane.

La Conferenza dei Capigruppo ha approvato il calendario dei lavori fino al 19 gennaio. Per la seduta odierna resta confermata la discussione dei disegni di legge di ratifica

si svolgerà il sindacato ispettivo e, alle ore 15, il *question time*, con la presenza dei Ministri della giustizia, dell'ambiente e della salute. In relazione alla richiesta di una informativa del Ministro degli affari esteri sui recenti fatti accaduti a Washington, è stato stabilito che questa avrà luogo presso le Commissioni congiunte affari esteri di Camera e Senato. L'Assemblea tornerà a riunirsi martedì 19 gennaio, alle ore 16,30, La Conferenza dei Capigruppo è convocata lo stesso giorno alle ore 15. I Capigruppo hanno, infine, convenuto di confermare, per la sessione annuale del 2021, senatori attualmente in carica nella delegazione parlamentare italiana presso l'Assemblea del Consiglio d'Europa.

adottata a Ginevra il 21 giugno 2019 nel corso della 108ª

ed altri. -*** ***Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro C 190 sull'eliminazione della violenza e delle molestie nel mondo del lavoro, fatta a Ginevra il 21 giugno 2019*** L'Assemblea è chiamata, quindi, all'esame di quest'atto, già approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati, e nel quale è stato assorbito l'Atto Senato 1598, di iniziativa parlamentare, recante la ratifica della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro n. 190 sull'eliminazione della violenza e delle molestie sul luogo di lavoro, adottata a Ginevra nel giugno 2019: quindi, recentissima. Si ricorda, innanzitutto, che la Convenzione sull'eliminazione della violenza e delle molestie nel mondo del lavoro è stata adottata a larga maggioranza nel corso della 108° sessione della Conferenza internazionale del lavoro il 21 giugno 2019, in occasione del centenario della creazione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), e che è frutto di un processo negoziale avviato nel 2015. Composto da 20 articoli, suddivisi in 8 titoli, il testo convenzionale rappresenta un importante strumento nell'azione di contrasto alle violenze e alle molestie commesse nel mondo del lavoro, con l'ambizioso obiettivo di proteggere tutti i lavoratori e tutte le lavoratrici a livello globale, a prescindere dal loro *status* contrattuale. La Convenzione fornisce, innanzitutto, una definizione piuttosto ampia, suscettibile di includere non soltanto l'abuso fisico, ma anche quello verbale, oltre a fenomeni di *stalking* e *mobbing*, di violenza e molestia, anche di genere, intesi come comportamenti e pratiche che provochino, mirino a provocare o siano suscettibili di provocare danni fisici, psicologici, sessuali o economici (articolo 1). Segnalo, altresì, che è in via di approvazione, da parte del Consiglio dell'Unione europea, la proposta di decisione COM(2020)24, che autorizza espressamente gli Stati membri a ratificare la Convenzione al nostro esame, in quanto alcune disposizioni del testo convenzionale sono contemplate dall'*acquis* dell'Unione nell'ambito della politica sociale e nel e nel settore della non discriminazione. In attesa della approvazione di tale proposta di decisione, alcuni Paesi, in particolare Francia, Belgio, Spagna e Svezia, oltre all'Italia, hanno già avviato la procedura di ratifica. di legge di ratifica si compone di quattro articoli. L'articolo 3, in particolare, pone una clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che, dall'attuazione della legge di ratifica, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Si delinea, quindi, un quadro solido e chiaro, normativamente e nell'individuazione delle definizioni delle varie forme di sfruttamento, disparità e discriminazioni.

(di paga, sono mobbizzate, sfruttate e violentate), o dove la vita di un bambino non vale nulla quando viene costretto a scavare nel fango in miniere o a raccogliere rifiuti tecnologici in enormi discariche. Noi abbiamo i tribunali, le leggi, le associazioni dei lavoratori. Loro non hanno nulla. Oggi è importante approvare questa Convenzione non solo per migliorare noi stessi, ma perché molti altri Paesi la ratificano. Signor Presidente, colleghi, non solo tra le pareti domestiche, ma sul lavoro una donna, un uomo, un bambino si possono far morire anche senza ucciderli. In conclusione, si propone l'approvazione del disegno di legge anche per loro.

Denise aveva diciannove anni quando è stata assunta in una società di spedizioni e ha iniziato a subire molestie dal suo datore di lavoro settantacinquenne, con *avance* che puntualmente ha rifiutato, nonostante nonostante fosse stata progressivamente demansionata e avesse subito anche peggioramenti contrattuali. Denise è stata più forte del suo aguzzino, ha trovato la forza di denunciare, ha scoperto che il suo datore di lavoro molestava anche una sua collega, di anni dalla denuncia, il tribunale di Pistoia ha stabilito la colpevolezza dell'uomo e un risarcimento per entrambe le dipendenti. È per le tante Denise in Italia che il voto di oggi assume una valenza anche etica. La Convenzione sull'eliminazione della violenza e delle molestie nel mondo del lavoro, adottata nel giugno scorso in occasione del centenario della creazione dell'Organizzazione internazionale del lavoro viene giustamente definita come una sentenza storica perché rappresenta un passo avanti concreto. Innanzitutto fornisce una definizione ampia di violenza e molestia: una definizione che include non soltanto l'abuso fisico ma anche quello verbale, oltre a fenomeni come lo *stalking* e il *mobbing*, perché fa espresso riferimento alle violenze e alle molestie fondate sul genere che possono provocare danni fisici, psicologici, sessuali sessuali ma anche economici. E poi si rivolge alla tutela di ogni lavoratore, indipendentemente dal fatto che sia dipendente o meno, a prescindere dal relativo *status* contrattuale. Si includono, quindi, anche i volontari, le persone nel corso di periodi di formazione, tirocinio e apprendistato, e arriva a tutelare anche coloro che sono alla ricerca di un lavoro o i lavoratori il cui rapporto sia stato addirittura estinto. Un'altra cosa positiva è che si riconoscono come violenze o molestie anche quelle che si verifichino al di fuori del posto di lavoro, inteso in senso fisico, ricomprendendo dunque tutte quelle condotte che si verifichino, ad esempio, durante viaggi di lavoro ed eventi sociali, così come nel contesto delle comunicazioni che avvengono per via telematica. Un aspetto rilevante, visto l'aumento di avvicinamenti o molestie legate al genere che avvengono sui nuovi *social* come WhatsApp, meno formali ma altrettanto insidiosi. La Convenzione, inoltre, prevede un articolato ventaglio di obblighi per gli Stati e, a seguire, anche per i datori di lavoro, che non sono più soltanto nella possibilità ma hanno il dovere di garantire garantire la tutela di tutti i soggetti nell'ambiente di lavoro. Quindi basta con gli atteggiamenti in cui si chiude un occhio o si fa un sorrisino. Con la ratifica di questa Convenzione, in sostanza, promuoviamo un rovesciamento dell'approccio culturale e dell'approccio collettivo al fenomeno. Si prevedono, tra l'altro, obblighi per i diversi Stati anche rispetto all'introduzione di poteri incisivi per gli ispettori del lavoro e delle altre autorità deputate al controllo. Oggi si stima che l'80 per cento delle donne che subiscono abusi dai propri colleghi di lavoro o dai propri responsabili, spesso non denunciano o non ne parlano proprio per quieto vivere o temendo scandali o ritorsioni. spesso queste violenze riguardano proprio chi è più precario all'interno del mondo del lavoro. Si tratta di un cambio, di una svolta. Non c'è atteggiamento goliardico che tenga. Si tratta di favorire una rivoluzione culturale che renda possibile un cambio di passo. Anche per questo è importante oggi ratificare questa Convenzione. Mi auguro che il voto possa vedere compatte le diverse forze politiche, a differenza di quanto avvenuto in Commissione, perché non si può parlare di ingerenze rispetto alla giurisprudenza nazionale. Quando si tratta di tutelare la dignità delle lavoratrici e dei lavoratori non ci devono essere motivazioni o scuse perché l'unica ingerenza è quella che tratta il corpo altrui come fosse un oggetto di sua proprietà, sul lavoro e fuori. Contro questo atteggiamento noi oggi andiamo a porre un argine. Ecco perché dichiaro convintamente il voto favorevole del Gruppo Italia Viva-PSI.

è organizzata in 20 articoli e divisa in 8 sezioni. Voglio però ricordare che sono trascorsi ben otto anni di dibattito prima che si arrivasse alla sua approvazione. Forse anche per questo tale approvazione è considerata, se non una data addirittura storica, sicuramente un importante spartiacque sul fronte dell'eliminazione delle violenze e delle molestie nel mondo e nei luoghi di lavoro e anche dell'opportunità di adottare nuove norme internazionali in materia. Un altro elemento distintivo che desidero sottolineare è l'approccio. Si tratta infatti di un approccio più ampio, ovvero si arriva alla conclusione che le violenze e le molestie sul luogo di lavoro riguardano tutti, uomini e donne,

la Convenzione ha un approccio che guarda a tutti, uomini e donne, anche se nella nota evidenza statistica che le donne sono colpite in modo maggiore e sproporzionato. La Convenzione e le sue norme internazionali sono anche il frutto di studi comparati delle leggi e delle pratiche nazionali in materia di violenza e molestie sul lavoro di ben 80 Paesi. Ci troviamo quindi di fronte a un quadro normativo internazionale estremamente articolato e complesso, con un'architettura molto salda. È importante

per cominciare. La raccomandazione n. 206, contestuale alla Convenzione, non ha evidentemente valore vincolante, ma è importante nella misura in cui contiene orientamenti su come applicare gli obblighi della suddetta Convenzione. Un altro elemento di riflessione: la Convenzione chiama in causa violenze e molestie nei luoghi di lavoro, ma porta con sé e cerca di dipanare anche una matassa complessa di temi e risvolti, come è stato già ricordato. Mi riferisco al al *mobbing*, allo *stalking*, alle violenze psicologiche, al tema della tutela dei lavoratori e a come prevenire e affrontare le violenze e le molestie. Vi è inoltre un passo ulteriore: si intende un'interpretazione ampia proprio perché si guarda a un insieme di comportamenti, pratiche e atti destinati a causare o anche minacciare un danno fisico, psicologico ed economico, o che si configuri - è previsto - come reato sessuale o come violenza di genere.

i corsi di formazione lavorativa lontani dal luogo abituale di lavoro, ma anche i mezzi di comunicazione e informazione come le *chat*, gli *sms*,le *e-mail*, i messaggi WhatsApp, cioè tutti quegli strumenti che, come sappiamo bene,

2016, in cui si affronta anche il capitolo delle violenze e delle molestie sul lavoro e dei ricatti sessuali. Richiamo solo un dato tra i tanti forniti dall'Istat: milioni sono le donne che nel corso della loro vita hanno subito molestie fisiche e ricatti sessuali sul posto di lavoro, ovvero l'8,9 per cento della forza lavoro femminile. La suddetta indagine rileva anche che nel triennio 2013-2016 a subire questi episodi sono state oltre 425.000 donne, ovvero il 2,7

contatti fisici subiti, richieste di prestazioni sessuali o disponibilità in cambio di promozioni o di concessione di un posto di lavoro oppure di un avanzamento, di una promozione o di fronte alla minaccia di licenziamento.

le molestie sui luoghi di lavoro che colpiscono donne e uomini; contro, punto e basta. Aggiungiamo solo un'ultima considerazione. Proprio perché tutto questo è importante, auspichiamo che non ci si limiti come Paese, come Nazione Italia a ratificare poi la Convenzione, ma a ma a seguirla nella sua applicazione, accompagnandola con una serie di provvedimenti che consolidino l'applicazione di questo principio, perché contestualmente dobbiamo aggredire anche altre questioni, come per esempio la disparità salariale a parità di lavoro svolto; dobbiamo consentire parità di accesso ai lavori e alle carriere anche alle donne; dobbiamo far sì che la maternità sia una libera scelta e non una scelta condizionata e potrei continuare, perché la materia è complessa. Termino davvero con una riflessione: cerchiamo di approfittare di questa occasione per rovesciare un antico pregiudizio che, come è noto, è qualcosa che precede il giudizio, che si basa sull'esperienza e la conoscenza. I pregiudizi sono un vizio della mente e noi auspichiamo che con questa opportunità si rovesci anche quel pregiudizio abituato a dare sempre queste colpe delle molestie al datore di lavoro e all'imprenditore. Le statistiche, infatti, ci rivelano che non è così: le molestie avvengono anche tra colleghi;

credo che oggi sia una giornata molto importante e francamente mi dispiace che l'Assemblea sia abbastanza distratta nel

internazionale del lavoro che impegna i Paesi ed è immediatamente operativa. È un impegno solenne che il nostro Paese sta assumendo andando ad approvare finalmente e a ratificare la Convenzione stessa. Rispetto ad altre convenzioni si è riusciti a farla approvare abbastanza

prima di me ricordava. L'indagine sulla violenza contro le donne condotta dall'Agenzia dell'Unione europea dice che una donna su due dichiara di aver subito una qualche forma di molestia sessuale cento dei casi il molestatore è un collega, un subalterno o un superiore e questi dati sono drammatici. Ancora più drammatici sono i dati dell'indagine Istat

di altro con cui si esercita un potere ricattatorio a sfondo sessuale. Nel momento del colloquio

Molto spesso il colloquio è accompagnato dal ricatto, dall'allusione e da un modo abbastanza per cento di questi ricatti viene ripetuto quotidianamente; viene ripetuto quotidianamente; il 17,4 all'incirca una volta a settimana; il 29,4 qualche volta al mese e il 19,2 più raramente. Ho voluto citare questi dati per dire

cento delle vittime intervistate non ne ha mai parlato e meno dell'1 per cento ha avuto poi il coraggio di denunciare quello che è accaduto oppure

abbiamo a disposizione un vero e proprio strumento nell'azione di contrasto alle violenze e alle molestie commesse nel mondo del lavoro, facciamo un atto fondamentale per sostenere le donne e chiunque subisca ricatti di questo genere sul posto di lavoro e soprattutto diamo loro la possibilità e la forza del rispetto della dignità. La Convenzione fornisce una definizione piuttosto ampia di molestia e violenza, in modo tale da coprire l'ampia gamma con cui questi elementi

L'ambito di applicazione è appunto la protezione delle lavoratrici e dei lavoratori, a prescindere - questo è fondamentale

gli obblighi agli Stati, quindi al nostro Stato, di adottare tutte le disposizioni interne che definiscano la violenza e le molestie e tutte le misure atte a prevenire queste condotte condotte lesive, anche dal punto di vista risarcitorio e repressivo. Ciò significa che richiede agli Stati di garantire alle potenziali vittime l'accesso alla giustizia in maniera effettiva, predisponendo misure atte a porvi rimedio.

per essere assunte o per mantenere il posto di lavoro. Se una donna subisce un ricatto sessuale, nell'80 per cento dei casi non ne parla con nessuno sul posto di lavoro; quasi nessuna fa denuncia,

queste ha cambiato volontariamente lavoro o ha rinunciato alla carriera a causa di ricatti sessuali sul luogo di lavoro; il 10 per cento è stato licenziato o messo in cassa integrazione. Questo è il quadro in cui l'Organizzazione internazionale del lavoro il 21 giugno 2019 adottava, con una larghissima maggioranza degli Stati membri, la Convenzione sull'eliminazione della violenza e delle molestie sui luoghi di lavoro. Il lavoro è il luogo dei diritti e dell'emancipazione delle persone e sono orgogliosa che l'Italia sarà il primo Paese tra i 187 membri a ratificare questa Convenzione. L'Italia è un Paese che già prevede norme antidiscriminatorie e a tutela dei lavoratori, ma oggi approviamo un quadro di riferimento e un programma di tutela decisamente innovativo. Mi preme sottolineare la natura internazionale di questo quadro normativo. Siamo ormai abituati ad associare alla parola «globalizzazione» la perdita dei diritti e il peggioramento delle condizioni di lavoro. Vogliamo ribaltare questa equazione e che ci sia una globalizzazione dei diritti contro lo sfruttamento delle persone,

Violenza e molestie sui luoghi di lavoro sono violazioni dei diritti umani e questo tipo di violenze, che si traduce in molestie fisiche, verbali e ricatti, purtroppo è ancora coperto da omertà, silenzi e mancanza di solidarietà, molto più che negli altri casi - già censurabili - di violenza. Come ho detto, quasi il 90 per cento delle donne che hanno subito non ha denunciato. È già stato detto dalle colleghe che mi hanno preceduto quali sono i principali contenuti innovativi. Innanzitutto, un ampliamento della definizione di violenza o di molestie, ma soprattutto del luogo: quello di lavoro non è soltanto il luogo fisico dello stabilimento, ma può essere anche

C'è un obbligo degli Stati membri di prescrivere e del datore di lavoro di adottare misure preventive e repressive e c'è l'obbligo di garantire l'accesso alla giustizia, nonché un maggiore coinvolgimento degli ispettori del lavoro. Il nostro Paese, in realtà, com'è stato detto, non arriva sguarnito su questo tema. Voglio ricordare due questioni per tutte: nella legge di bilancio del 2018 abbiamo introdotto il divieto di demansionamento, licenziamento e trasferimento a seguito di denuncia di molestie sessuali, nonché la nullità del licenziamento ritorsivo o del demansionamento della persona denunciante,

della collega Fedeli e della collega Valente aventi proprio a oggetto i temi della tutela e dell'antidiscriminazione sui luoghi di lavoro. di lavoro. Molestie e ricatti sessuali affondano le radici in modelli culturali, quindi è di nuovo la scuola il principale campo di contrasto sul quale sempre dobbiamo investire e impegnarci per una diversa consapevolezza e appartenenza a modelli culturali. La causa principale sta però nello squilibrio di potere tra chi agisce la violenza e chi la subisce. Voglio ricordare le parole di Guy Ryder, direttore generale dell'OIL, quando dice che bisogna mettere in pratica questi diritti al fine di creare un ambiente lavorativo migliore, più sicuro e dignitoso per donne e uomini. Voglio concludere con un'ultimissima riflessione. Parliamo

e riscatto delle persone, perché segna il rapporto tra la persona e la collettività ed è anche e soprattutto da questo che passa l'essere cittadini e non sudditi.

per legiferare su questi temi e attuare pienamente la Costituzione. Governo, onorevoli colleghi, vorrei anzitutto ringraziare per la relazione esaustiva il collega Airola e le colleghe che mi hanno preceduto per gli appassionati interventi su un tema così delicato, che riscalda la sensibilità di ciascuno di noi. Infatti, credo che sia un principio di civiltà quello che stiamo difendendo

La ratifica della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro per l'eliminazione della violenza e delle molestie sul luogo di lavoro che stiamo per approvare trova tuttavia, di fatto, già pieno riconoscimento nel nostro ordinamento. Ricordo che nel 2006,

e opportunità tra donne e uomini in tutti i campi, compresi l'occupazione, il lavoro e il trattamento economico. L'articolo 26 del citato codice ha sancito, tra l'altro, un'equiparazione tra molestie sessuali e discriminazione di genere. La legge di bilancio, per il triennio 2018-2020, modificando il suddetto articolo 26, ha previsto inoltre una specifica tutela per chi agisce in giudizio per aver subito, appunto, una molestia sessuale sul luogo di lavoro.

Certamente il Parlamento non considera esaurito il proprio ruolo riguardo a temi così importanti, come quello della parità di trattamento senza distinzione di genere della concreta rimozione degli ostacoli per consentire a qualsiasi individuo la piena partecipazione alla vita economica, politica e sociale del nostro Paese.

dall'Organizzazione internazionale del lavoro il 21 giugno 2019, con l'obiettivo di eliminare la violenza e le molestie nel mondo del lavoro. È importante chiarire che, come Gruppo, condividiamo i nobili obiettivi della Convenzione, perché sradicare il problema delle molestie e della violenza di ogni genere dai luoghi di lavoro dev'essere un obiettivo primario per un Paese civile. L'importanza del tema del lavoro è il faro della nostra attività politica. Un Paese sano è un Paese che lavora per questo, ogni attenzione che possa migliorare la tutela dei lavoratori nel proprio ambiente di lavoro è un obiettivo da perseguire. Questo però non ci preclude la possibilità, come abbiamo fatto anche in Commissione, di esprimere alcuni dubbi sugli effetti che potrebbero avere sull'Italia le modalità di applicazione della Convenzione all'interno del nostro ordinamento, al momento non del tutto chiare. Il testo prevede infatti un articolato quadro di obblighi per gli Stati membri, a partire da quello di adottare disposizioni interne che definiscano le violenze e le molestie conformemente a quanto previsto dalla Convenzione e che prescrivano ai datori di lavoro di porre in essere tutte le misure atte a prevenire le condotte lesive, fino al più generale obbligo per gli stessi Stati di adottare le misure necessarie, sia preventive sia repressive. La Convenzione sarà poi soggetta al meccanismo di controllo previsto dall'Organizzazione internazionale del lavoro, anzitutto attraverso i rapporti periodici presentati dagli Stati. È previsto inoltre un meccanismo speciale, che consente a uno Stato membro di presentare all'Organizzazione una denuncia nei confronti di un altro Stato che non abbia assicurato l'efficace attuazione della Convenzione stessa. Mi chiedo, quindi, cari colleghi, se non vi sia il rischio di aprire un nuovo terreno di conflitto tra Stati, che si basa su lotte di natura giudiziaria, che nascondono invece vere e proprie volontà di attaccare, sul piano internazionale, un Paese o un Governo non gradito. inoltre considerato anche il potere di denuncia che viene riconosciuto al consiglio d'amministrazione della stessa Organizzazione e perfino ai singoli delegati presso la Conferenza internazionale del lavoro, rendendo possibile l'attivazione, su loro iniziativa, di una procedura passibile di condurre alla creazione di una Commissione d'inchiesta, incaricata di redigere un rapporto contenente, eventualmente, anche raccomandazioni per lo Stato interessato. La controversia potrà sfociare anche in un giudizio della Corte internazionale di giustizia, aprendo quindi la via una nuova compressione della sovranità nazionale del nostro Paese. Signor Presidente, in conclusione, non mancano quindi elementi di perplessità, che ho tenuto ad esprimere e condividere con i colleghi. Come già ripetuto in premessa, non siamo contrari ai principi che la Convenzione promuove, ma abbiamo dubbi sulla loro traduzione in pratica. Nonostante questi elementi di incertezza, visti gli obiettivi condivisibili di questa Convenzione, esprimo il voto favorevole del Gruppo Lega-Salvini Premier-Partito

quando un'eco lontana e un po' confusa del grande movimento femminile Me Too arrivò anche qui da noi in Italia, in Italia, la reazione del nostro Paese non mi rese particolarmente orgogliosa. Si preferì infatti perdersi dietro al *gossip* e al voyeurismo e mettersi a sindacare se quella attrice o quell'altra fossero effettivamente degne di credito, finendo così per andare dietro a casarecci processi mediatici nei *talk show* o sui rotocalchi, anziché mettere a fuoco il problema e il suo impatto. Tale impatto è a dir poco sconcertante. Molestie, violenze e ricatti sessuali sul luogo di lavoro: quante donne ne sono vittime? È persino difficile stimarlo, perché non esiste una specifica fattispecie di reato e non c'è mai stato un monitoraggio regolare e costante di questo tipo di violenza. Per farcene un'idea, dobbiamo ricorrere all'unica indagine Istat esistente, che risale al 2016. I dati emersi sono preoccupanti: infatti, sono 1,404 milioni le donne che, nel corso della loro vita lavorativa, hanno subito molestie fisiche o ricatti sessuali sul posto di lavoro. Rappresentano l'8,9 per cento delle lavoratrici, ivi incluse le donne in cerca di occupazione. Parliamo quindi di una donna su dieci. Limitatamente ai ricatti sessuali sul lavoro, sono invece 1,173 milioni, il 7,5 le donne che, nel corso della loro vita lavorativa, sono state sottoposte a qualche tipo di ricatto sessuale per ottenere un lavoro, mantenerlo o ottenere progressioni nella loro carriera. Non è tutto, il termometro migliore per avere il polso della situazione consiste in un altro dato, ossia che, nell'81 per cento dei casi, la donna vittima di tali comportamenti non ne parla con nessuno sul posto di lavoro. Per non parlare delle denunce: solo lo 0,7 per cento delle vittime di ricatti ha sporto denuncia alle forze dell'ordine. Perché, di fronte a un fenomeno tanto vasto, le denunce sono invece così poche? Per ragioni piuttosto ovvie: la paura di non essere credute o di essere addirittura colpevolizzate, di perdere il posto o che tutto sia vano. Possiamo dare loro torto? Direi di no. Basti pensare al caso eclatante avvenuto l'estate scorsa, quando il presidente della società di trasporti lucana, la Cotrab, pur essendo stato processato e condannato con sentenza definitiva a due anni e sei mesi per violenza sessuale ai danni di una dipendente, è stato poi rieletto dagli stessi consorziati. Quella donna rientrava in quello 0,7 per cento delle vittime che trovano il coraggio di denunciare, sfidano la paura di perdere il posto di lavoro e di non essere credute e affrontano un lungo processo. Il colpevole viene condannato, ma poi tutto rischia di essere vanificato da una subcultura che normalizza e banalizza la violenza sessuale sul lavoro. Per fortuna, ci ha pensato l'ondata di indignazione generale a ripristinare davvero la giustizia, convincendo il colpevole a dimettersi. L'episodio dimostra che gli strumenti attuali non sono sufficienti a contrastare quest'odioso fenomeno. Mi sento di sottoscrivere la preoccupazione manifestata, tra gli altri, dalla Fondazione studi consulenti del lavoro, che sottolinea come gli effetti nefasti della pandemia da Covid-19 sull'occupazione femminile, quali l'accresciuta precarizzazione lavorativa e il conseguente disagio economico e sociale, possano contribuire ad aggravare ulteriormente il fenomeno delle molestie e soprattutto dei ricatti sul luogo di lavoro. Ricordo che già nel 2019 la Commissione femminicidio - di cui mi onoro di far parte - aveva dedicato il 25 novembre di quell'anno proprio al contrasto alla violenza e alle molestie sul luogo di lavoro, sottolineando come il lavoro sia un diritto universalmente riconosciuto e come, tuttavia, proprio il lavoro rappresenti purtroppo ancora un luogo di disparità tra uomini e donne. Salutiamo quindi con favore il traguardo dell'odierna ratifica della Convenzione dell'OIL, che sancisce che violenza e molestie costituiscono una violazione o un abuso dei diritti umani e riconosce il diritto di tutti e tutte a un mondo del lavoro libero da violenza e molestie.

Ci sono disegni di legge depositati da diverse colleghe, tanto di maggioranza quanto di opposizione, per normare questa specifica fattispecie di reato, violenza e molestie sui luoghi di lavoro: mi auguro che se ne possa iniziare presto l'esame. Ricordo peraltro, sommessamente, che anche le Forze armate costituiscono un luogo di lavoro. Le donne sono entrate a farne parte da ormai ventun anni; non è più possibile quindi procrastinare, a questo punto, l'introduzione, anche all'interno del codice militare penale, dello specifico reato di violenza e molestie sessuali. Anche in questo caso, vi sono disegni di legge in materia che attendono di essere approvati, tra i quali uno specifico a mia prima firma. Speriamo di non dover sentire mai più - né fuori né dentro quest'Aula - che, se una donna è oggetto di attenzioni sessuali non richieste, è perché lei è provocante, non perché lui è un molestatore che, se una donna ha ottenuto un posto di lavoro o una promozione, è perché si è concessa alle persone giuste. Rimettiamo l'inquadratura nel verso giusto e impariamo a distinguere chi sono le vittime e chi gli aguzzini.

***Ratifica ed esecuzione dello Scambio di note di modifica della Convenzione del 19 marzo 1986 per la pesca nelle acque italo-svizzere tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera, fatto a Roma il 10 e il 24 aprile 2017***

ed esecuzione dello scambio di note, sottoscritto dall'Italia e dalla Confederazione elvetica nell'aprile 2017, per la modifica della Convenzione bilaterale risalente al 1986, relativa, appunto, alla pesca nelle acque italo-svizzere. Ricordo innanzitutto che la Convenzione bilaterale del 1986 è lo strumento normativo che la Svizzera e l'Italia hanno sottoscritto al fine di assicurare la gestione ottimale ottimale del patrimonio ittico delle acque italo-svizzero dei laghi Maggiore, di Lugano e del fiume Tresa e, in particolare, per favorire lo sviluppo delle categorie che operano nel settore della pesca professionale e dell'attività di pesca sportiva, nonché per contribuire alla difesa e al miglioramento dell'ambiente acquatico. Lo scambio di note in esame reca una modifica della Convenzione al fine di adeguarla alle mutate situazioni ambientali, all'accresciuto corpo di conoscenze scientifiche, all'emergere di nuove problematiche e all'esigenza di rendere più agile l'ordinamento previsto dalla Convenzione medesima. Il disegno di legge di ratifica si compone di quattro articoli. In particolare, l'articolo 3, emendato a seguito del parere formulato dalla Commissione bilancio, pone una clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che per le attività derivanti dallo scambio di note si provveda con le risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che le amministrazioni competenti diano attuazione alla legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili. Il provvedimento non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento dell'Unione europea e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese. In conclusione, si propone l'approvazione del disegno di legge da parte dell'Assemblea del

esame riguarda il Protocollo n. 15 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo che ha istituito la Corte di Strasburgo nel 1959,

membri, in conformità al principio di sussidiarietà, hanno la possibilità di intervenire con un apprezzamento e un maggior margine di azione nell'attuazione delle disposizioni della Convenzione, sempre sotto il controllo della Corte.

il processo, riducendo - ad esempio - da sei a quattro mesi il periodo di tempo in cui si può adire la Corte europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

modo viene modificata in parte la condizione di ricevibilità di un ricorso, ampliando il margine della Corte sull'entità del pregiudizio subito dal ricorrente. Il disegno di legge prevede solo tre articoli, riguardanti l'autorizzazione alla ratifica, l'ordine di esecuzione e l'entrata in vigore del provvedimento. Non ci sono oneri per la finanza pubblica non ci sono profili di incompatibilità con la normativa nazionale, con l'ordinamento europeo e con gli obblighi internazionali. In conclusione, si propone l'approvazione del disegno di legge da parte dell'Assemblea

della Corte, ossia il principio che anche la giurisdizione nazionale si può occupare - e ci mancherebbe altro - di garantire il rispetto dei diritti e delle libertà definiti nella Convenzione,

sovverte tutta la giurisprudenza costituzionale italiana emanata fino a oggi. Ricordo che la giurisdizione italiana è sovrana

della Corte europea. E ciò non ci convince per numerose ragioni di ordine costituzionale, ma anche di ordine politico.

a importanti magistrati, a cominciare da Falcone e Borsellino; misure depotenziate da una pronuncia della Corte europea che a parole ha scandalizzato tutti - salvo oggi la maggioranza che vota - e che ci sottopongono ulteriormente al suo controllo. L'articolo depotenziato dalla pronuncia della Corte europea, è il frutto di sacrifici di intere generazioni, che è stato fondamentale per combattere la criminalità e la mafia nel nostro Paese. lo ha messo in discussione e noi, anziché contestare questo, gli diamo ancora maggiore controllo sull'attività giurisdizionale italiana. Non è solo questo il punto:

dai principi che la Corte europea dei diritti dell'uomo vuole imporre agli Stati membri appartenenti alla Convenzione, in ossequio a un'ideologia che viene

e di cultura latina come l'Italia. Per queste ragioni noi non siamo d'accordo a inginocchiarci ulteriormente a questi principi e per tale ragione dichiariamo convintamente il nostro voto contrario.

che potrebbero ledere l'autonomia della giurisdizione nazionale - criticità peraltro già emerse in prima lettura alla Camera nel dibattito che si è svolto

Signor Presidente, colleghi, membri del Governo, annuncio in maniera molto

fin dalla scorsa legislatura e continuo a farlo adesso. Le cose cambiano e magari cambieranno anche in futuro ma non lo so. Continuerò in ogni caso a votare conformemente in questo modo su atti di siffatto tipo.

sovranazionale, soprattutto in campo giuridico, su temi che sono invece prettamente nostri, prettamente intimi alla nostra giurisdizione. Siamo fortemente preoccupati per alcune

Signor Presidente, invito veramente i colleghi a ripensare

CEDU è un atto sbagliato e gravissimo. La CEDU ha indebolito e ha messo in discussione i capisaldi della lotta alla mafia; ha dimostrato gravissime lacune nella conoscenza dello stesso ordinamento italiano, quando lo ha confuso con un ordinamento di *common law* nella famosa e disgraziata sentenza Contrada, ritenendo erroneamente che il diritto penale fosse di creazione giurisprudenziale; cosa che, se venisse ripetuta in un'aula universitaria, comporterebbe l'immediata fine dell'esame del povero studente. ora ribadire in un trattato che i nostri giudici devono essere sottoposti al controllo di siffatto organismo, le cui lacune sono state evidenziate

Siamo in un momento sicuramente critico della vita di questa legislatura. Ci sono venti di tempesta che si accumulano e c'è una posizione che io credo credo testimoni più di ogni altra come questo Governo non sia stato all'altezza delle aspettative dei suoi parlamentari. Mi riferisco, concretamente, al rapporto che c'è tra le interrogazioni presentate e le risposte ricevute.

Ho presentato 41 interrogazioni a risposta orale e ho ricevuto 6 risposte; ho presentato 64 interrogazioni a risposta scritta, pensando che fosse più facile ottenere una risposta, e ancora una volta ho ottenuto 6 risposte, corrisponde a meno del 10 per cento di tutte le domande fatte e di tutti i quesiti posti. Se teniamo conto che le interrogazioni sono uno degli strumenti più importanti con cui il singolo parlamentare porta all'attenzione del Ministro un problema emerso sul territorio, nella vita di un'associazione, nella vita di una persona, questo dà l'idea del profondo disinteresse con cui da parte del Governo ci si è fatti carico di una delle manifestazioni più tipiche del lavoro del parlamentare. Sollecito quindi le risposte

per ottenere le risposte, ma è lo stile di lavoro ad essere veramente indecente. Non è possibile che un parlamentare si faccia carico delle istanze del suo territorio per portarle all'attenzione del Governo e quest'ultimo non consideri in alcun modo questo come un punto qualificante del suo lavoro. Penso che molti colleghi sappiano che a Londra, nel Parlamento, il Governo è tenuto a rispondere nell'arco di due settimane.

Signor Presidente, nel commemorare l'intellettuale Leonardo Sciascia in occasione del centenario della sua nascita, non posso celare l'ammirazione e l'affetto che provo davanti a una personalità così eccelsa. Credo così di interpretare anche il pensiero di molti colleghi siciliani presenti in Aula, in omaggio alla nostra "sicilitudine", come la chiamava lui. Leonardo Sciascia: un grande intellettuale siciliano purtroppo poco compreso in vita, che non smette però di essere fonte illuminante e guida anche nei nostri giorni. La sua antiveggenza lo ha esposto a feroci critiche e solo il tempo l'ha reso comprensibile ai più, anche da parte di chi all'epoca si è sentito direttamente colpito, soprattutto comprendendo che la sua attività di scrittore era contigua a quella di giornalista. È stato l'estrema propaggine in terra di Sicilia del pensiero illuminista; indagatore irrequieto e soprattutto attento al recupero del contesto, come gli insegnò il suo autore preferito, Alessandro Manzoni. Dell'intellettuale illuminista lui ebbe la fiducia, l'analisi condotta alla propria maniera con un'amara ironia; un intento che seppe declinare in mille varianti nelle sue opere e nei suoi articoli e avente come scopo sempre l'utile. un intellettuale di cui oggi si sente una profonda mancanza e necessità, lontano dal conformismo e da ogni compromesso, nonché scevro da ogni cortigianeria. Sciascia ci racconta fatti che non sono mai ciò che sono o quantomeno non sono solo quello: sono metafore, apologhi per comprendere ben altro. Parlare di mafia in tempi in cui se ne negava l'esistenza e coglierne la capacità trasformista e mimetica all'interno della società è stata veramente un'intuizione straordinaria, considerati i tempi in cui fu pubblicato «Il giorno della civetta»,

politica, popolarità e antimafia, in cui spiegò come l'antimafia può diventare un formidabile strumento per fare carriera, procurarsi il consenso del pubblico e acquisire crediti. Di ciò Sciascia fa anche una sorta di archeologia, partendo da lontano e precisamente dall'operato del prefetto Mori, mandato in Sicilia dal Governo fascista per risolvere *manu militari* la questione, che gli valse l'avanzamento della carriera. Arrivò poi ai suoi giorni, svelando la pericolosità insita nell'antimafia, di cui quella più grave è ricorrere a essa per avere poteri straordinari e momentanea sospensione dello Stato di diritto. Per Sciascia la vera sfida era vincere la mafia con strumenti ordinari, senza indulgere a derive autoritarie o deliri di onnipotenza. Il suo auspicio, che faccio mio, è che in un'epoca come la nostra, caratterizzata dalla straordinarietà, si possa ristabilire al più presto un clima di normalità e che soltanto con una vittoria morale che ci coinvolgerà tutti a livello sia individuale, che istituzionale si potrà vincere la mafia e non certo - e non solo - con l'autoritarismo. Signor Presidente, onorevoli colleghi, voglio esprimere a nome mio e di tutta l'Assemblea la piena solidarietà e vicinanza al sindaco di Pomigliano d'Arco, professor Gianluca Del Mastro, per il vile atto intimidatorio che ha ricevuto. La busta recapitata, contenente all'interno un proiettile insieme a una lettera intimidatoria nella quale gli si chiede di dimettersi per il suo bene, rappresenta un atto di violenza che ha la stessa valenza di un'aggressione fisica personale. Ovviamente rispettiamo il lavoro di indagine che le Forze dell'ordine stanno svolgendo. Molto spesso accade che chi svolge un ruolo nell'interesse della comunità sia oggetto di pressioni e atti minatori, perché la strada della legalità, della trasparenza e del rinnovamento è un percorso difficile, costellato di insidie e ostacoli. Ma chi opera nell'interesse dei cittadini e della collettività non ha e non deve avere timore ed è per così dire vaccinato rispetto a episodi di vigliacca arroganza. la mia piena solidarietà al sindaco Del Mastro, che invito a proseguire la sua attività istituzionale a testa alta. *(Applausi)*. Signor Presidente, gentili colleghi, vorrei chiedere la vostra attenzione su un fatto di rilevanza nazionale verificatosi giovedì scorso nella mia città di elezione, Ferrara. Parlo della lettera offensiva giunta al Museo nazionale dell'ebraismo italiano e della Shoah (MEIS). Al di là della fiducia dovuta all'operato delle Forze dell'ordine, che stanno indagando per comprendere se si tratta dell'azione isolata di un singolo oppure se rientra in un quadro più complesso, credo non si possa non esprimere non solo sdegno, ma anche preoccupazione. In un caso come nell'altro si conferma che nel 2021 continua a serpeggiare e germogliare odio, di cui gli ebrei sono da sempre facili bersagli. Il MEIS produce iniziative di grande interesse e lo ha fatto anche nel 2020, un anno difficile, promuovendo rassegne in remoto atte a diffondere la conoscenza della cultura ebraica in Italia. Non ha sospeso la propria attività, tutt'altro. La missiva al MEIS, fosse stata inviata anche da un balordo, ha dunque un preciso significato; la destinazione è non casuale, ma precisa, sono le offese contenute. Va detto che a Ferrara c'è una storica comunità ebraica, perfettamente inserita, con cui esiste un dialogo profondo, intenso e continuativo a tutti i livelli istituzionali. Ferrara è la città in cui la nostra senatrice Liliana Segre è venuta, 2019, incantando una platea di 700 studenti in un teatro gremito, raccontando la sua esperienza di sopravvissuta ad Auschwitz. Ed è la città in cui l'amministrazione, oggi a conduzione leghista, le ha voluto concedere nello stesso anno la cittadinanza onoraria, per il profondo legame, intessuto nel tempo. Ferrara è la città di Bassani, dei Finzi Contini e la città del MEIS. Fatto non trascurabile è che la missiva è stata inviata nell'approssimarsi della Giornata della memoria, il 27 gennaio, ricorrenza dedicata alle vittime dell'Olocausto, nel ricordo dell'apertura,

immagini di Hitler, insulti del tipo «Ebrei ai forni», «Vi bruceremo tutti», e mi fermo qui. Si tratta quindi di un attacco scientificamente organizzato, sfruttando i nuovi strumenti digitali. Difficile pensare a una casualità, soprattutto nel momento in cui spinte neonaziste si stanno risvegliando ovunque in Europa. Cito ad esempio la Germania e non solo. All'attacco di Capitol Hill, lo scorso mercoledì notte, c'erano gruppi neonazisti. Stiamo assistendo a una recrudescenza dell'odio, fenomeno tipico nei momenti di disagio e di malessere sociale, quando le ideologie attecchiscono con più facilità, perché affondano e si cementano nell'insoddisfazione e nella frustrazione della gente, cui viene presentato un nemico per favorire la lotta dell'uno contro l'altro. Se gli ebrei da sempre - come dicevo poco fa - sono bersaglio facile, la crisi pandemica che stiamo vivendo è terreno fertile per coltivare e instillare ulteriori paure. Chiedo dunque l'impegno di tutti i presenti a monitorare, presidiare e a prendere le distanze da simili episodi, che non possono essere derubricati come minori, solo perché non hanno effetti devastanti, perché non è così: tra gli effetti c'è il rischio dell'emulazione che generano. Alla fiducia nelle Forze dell'ordine va accompagnata una costante campagna di sensibilizzazione. Concludo il mio intervento ricordando, doverosamente, le parole del presidente del MEIS e del direttore: «L'atto ignobile e vigliacco non fa che aumentare la determinazione e la tenacia con cui il museo conduce e condurrà la missione assegnatagli assegnatagli dal Parlamento italiano di tenere viva la memoria, di lottare contro l'antisemitismo ed educare le nuove generazioni ai principi di eguaglianza e fratellanza che la nostra Costituzione ci chiama a perseguire». *(Applausi)*.

la parte terminale della lavorazione, del riciclo, della differenziazione del rifiuto delle automobili. Si tratta, in parole povere, di parti in tessuto, gommapiuma,

europei gli scarti provenienti dalla trasformazione del petrolio vengono ridotti al minimo, in quanto sono utilizzati come combustibili, per l'alto valore energetico. Pertanto, auspico che in Italia si arrivi alla medesima soluzione, rendendo inutili o riducendo il volume delle relative discariche. Voglio infatti parlare di una discarica. A Verona, in quel di Sorgà, in località De Morta, è stata presentata la richiesta, nei confronti della Regione Veneto, di realizzare una discarica, che occupa una superficie complessiva, nel progetto, di 455.000 metri quadrati.

non trovando alcun tipo di risposta. Il Comune di Concamarise, in provincia di Verona, nel quale sono onorato di svolgere la carica di sindaco, ha espresso il suo no, come riportato nel quotidiano «L'Arena» del giorno 11 febbraio 2020.

una pianificazione a livello nazionale. Ci sono gli incentivi per le auto a livello fiscale (auto elettriche e auto ibride, con rientro dell'usato), che fanno sì che si aumenti solo questo tipo questo tipo di rifiuto, che non ha alcuna altra possibilità se non finire in discarica. Pertanto, il problema va risolto a monte, e non a valle, sui territori regionali.